L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. sono in corso i lavori della Conferenza dei Capigruppo. Sospendo pertanto la seduta fino alla conclusione della stessa. (La seduta, sospesa

la Conferenza dei Capigruppo ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 21 dicembre. L’ordine del giorno della seduta odierna è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni. La seduta di domani sarà dedicata al sindacato ispettivo e al question time, con la presenza dei ministri Di Maio, Bonafede e Tria. Martedì 27 novembre, con seduta dalle ore 9 fino alle ore 21, sarà discusso il decreto-legge in materia fiscale. Il calendario della prossima settimana prevede, inoltre, la discussione di mozioni contro la violenza sulle donne, il disegno di legge di delega al Governo per l’adozione di decreti correttivi di crisi d’impresa, la legge europea 2018 con le connesse relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e, inoltre, comunicazioni del Governo sulle decisioni in materia di bilancio. Martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 15, saranno discussi, fino alla loro conclusione, il rendiconto e il bilancio interno del Senato. Nelle sedute successive, fino - se necessario - a venerdì 7 dicembre, è prevista, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, la discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il disegno di legge collegato sulla pubblica amministrazione, nonché le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge di bilancio. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio, per la quale è stato definito un calendario di massima che prevede la conclusione dell’esame del disegno di legge di bilancio presumibilmente entro la giornata di venerdì 21 dicembre. Nella settimana dal 10 al 14 dicembre, che sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio, l’Assemblea potrà riunirsi per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, nonché per l’esame del disegno di legge anticorruzione - ove trasmesso dalla Camera dei deputati - e del disegno di legge di ratifica sulla Convenzione di Faro sul patrimonio culturale, ove concluso dalla Commissione. Infine, nelle settimane del 26-29 novembre e del 4-7 dicembre si terranno sedute di sindacato ispettivo e, alle ore 15 del giovedì, il question time. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 920 recante: «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo», Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5[a] Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

«La Commissione programmazione economi- ca, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall’articolo 10, comma 6, della legge di contabilità». Ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 920 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.